Comunico che in data 14 aprile 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie:* «Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche». Comunico che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea i senatori Raffaele De Rosa, Francesco Giacobbe, Roberto Menia ed Elena Murelli. Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Delegazione i deputati Salvatore Caiata, Isabella De Monte e Roberto Pella. D'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'INCE è convocata per mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 9,

Nella seduta di oggi sarà anticipata la discussione del decreto-legge per la protezione delle persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati. L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione delle questioni pregiudiziali, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, sul decreto-legge immigrazione e la trattazione nel merito del provvedimento stesso. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 19,30 di oggi. Il calendario della settimana, fermi restando gli altri argomenti già previsti, è integrato con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione. Giovedì 20 aprile, alle ore 15, avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri degli affari esteri, della giustizia e per lo sport. Il calendario dei lavori della prossima settimana, a partire da mercoledì 26 aprile, alle ore 12, è integrato con un'informativa del ministro Fitto sullo stato di attuazione del PNRR e con l'esame del DEF 2023 e dell'annessa Relazione, per la quale è necessario il voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Il previsto *question time* non avrà luogo.

Signor Presidente, cari colleghi, il disegno di legge in esame, n. 632, ha ad oggetto la conversione del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2023. Esso si compone di 6 articoli. L'articolo 1 dispone la proroga - fino al 31 dicembre 2023 - delle attività di assistenza e accoglienza già autorizzate il decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea a causa della crisi ucraina. Tra queste, è contemplata la prosecuzione delle forme di accoglienza diffusa nei limiti di 7.000 posti tramite convenzioni territoriali tra Regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile. Si dispone altresì la prosecuzione delle forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari di protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, nonché un incremento del contributo forfettario *una tantum* per l'ampliamento dei servizi sociali offerti dai Comuni che ospitano un significativo numero di soggetti richiedenti permesso di protezione temporanea. Difatti, a seguito di un intervento emendativo della Camera, il Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno è autorizzato a procedere al trasferimento *pro quota* delle predette risorse in favore dei Comuni beneficiari sulla base delle risultanze di un censimento aggiornato. Per lo stesso fine di garantire la continuità della gestione emergenziale, il comma 2 dell'articolo 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile a disporre, con proprie ordinanze, la rimodulazione delle misure in questione ai sensi dell'articolo 25 del codice della Protezione civile. Il comma 3 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure in parola nel Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della Protezione civile. I commi 4 e 5 dispongono degli incrementi di spesa per l'anno 2023, volti ad assicurare il potenziamento delle strutture di prima accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, nonché delle politiche e dei servizi dell'asilo. Infine, il comma 6 attribuisce al Ministero della salute, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'onere di verificare, entro il 30 aprile 2023, i costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché di estendere il godimento in favore dei profughi ucraini a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani fino al 31 dicembre del 2023. L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca la proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina fino al 31 dicembre 2023. L'articolo 2 inerisce invece ai permessi di soggiorno già rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea, con scadenza al 4 marzo, in adesione alla decisione di esecuzione n. 382 del 2022 del Consiglio dell'Unione europea. Di tali permessi di soggiorno è ammessa una proroga fino al 31 dicembre 2023, fatta salva la possibilità di sopravvenuta inefficacia o revoca nel caso in cui il medesimo Consiglio decida per la cessazione della protezione temporanea. L'articolo 2-*bis*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera, proroga, sempre fino al 31 dicembre 2023, la possibilità, riconosciuta ai professionisti residenti in Ucraina, di esercitare temporaneamente la professione sanitaria o la professione di operatore sociosanitario all'interno del territorio italiano, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private. L'articolo 3, intervenendo sull'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, istituisce un contributo, in luogo del precedente rimborso, in favore dei Comuni ospitanti minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, fermo rimanendo l'importo massimo di 100 euro al giorno *pro capite*. Si identifica inoltre il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno come struttura di supporto incaricata della gestione dell'emergenza in parola. I Comuni interessati a ottenere il contributo testé indicato sono tenuti a presentare istanza entro il 31 settembre 2024. Proprio in ragione dell'elevato numero di richieste di protezione internazionale derivante dal conflitto bellico, l'articolo 4 autorizza la Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, di non più dieci unità di lavoratori con contratto a tempo determinato che siano in possesso dei requisiti professionali necessari. L'articolo 5 dispone un incremento del Fondo per le emergenze nazionali pari a 61,5 milioni di euro per il 2023 e ne contempla la conseguente copertura finanziaria. Infine, l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

era il 24 febbraio dello scorso anno quando la Russia dava il via all'aggressione dell'Ucraina con dispiegamento di uomini e mezzi ingente. Da quel momento, Presidente, in tutta la Nazione si vive sotto le bombe, bersaglio dei missili russi e della ferocia dei battaglioni, che poco a poco hanno invaso quel territorio. La stragrande maggioranza della comunità internazionale non ha mancato di stigmatizzare l'accaduto ed ha preso immediatamente le distanze dalla politica russa. Con un attivismo senza precedenti, rapidamente, l'Unione europea ha messo in campo una serie di pacchetti sanzionatori nei confronti della Federazione Russa che iniziano a dare i loro frutti. Si pensava che la *leadership* energetica della Russia avrebbe potuto schiacciare l'Europa sotto il peso della mancanza di approvvigionamenti, ma sin da subito l'Europa si è adattata al nuovo scenario internazionale, facendo fronte alle esigenze energetiche delle popolazioni. Di più,

sono state inviate armi di difesa, armi tattiche, dispositivi moderni utili a respingere i costanti e pesantissimi attacchi aerei. L'Italia ha fatto e sta facendo la propria parte. I nostri militari, cui - non dimentichiamolo mai va tutta la nostra riconoscenza, si stanno adoperando in uno sforzo encomiabile per poter inviare a Kiev quanto loro necessita. In questo scenario, accanto alla distruzione sistematica delle infrastrutture ucraine, emerge un altro problema di fondamentale importanza, che è costituito dall'esodo massiccio del popolo ucraino verso l'Europa e naturalmente quota parte verso la nostra Nazione. Il Consiglio europeo ci informa che al 31 dicembre 2022 i rifugiati ucraini ospiti nelle nostre Nazioni ammontavano a 4,8 milioni e adesso hanno superato i 5 milioni. Unite per i rifugiati (UNHCR), i profughi che hanno richiesto protezione temporanea sono 173.213. Per dare un'idea, in Germania sono 900.000; di tutta evidenza, signor Presidente, che l'Italia è chiamata a dare il proprio contributo in ragione della solidarietà umana che nei secoli ha sempre mostrato nei confronti di chiunque, realmente bisognoso, abbia varcato i nostri confini. Su questo solco, il decreto-legge di cui oggi ci occupiamo indica con chiarezza e coerenza politica, l'accoglienza da parte del Governo, che non può che vedermi concorde sia nell'approccio che nel metodo.

Dell'aiuto ai popoli oppressi da una guerra ingiusta e subita, noi, l'Europa, dobbiamo fare la nostra bandiera, fermo restando che la vigilanza delle frontiere deve restare altissima. In questo senso desidero rivolgere una raccomandazione al Governo. I flussi migratori derivanti da conflitti portano con sé molti autentici profughi, ma purtroppo anche organizzazioni dedite al crimine che, sull'onda lunga della solidarietà, si insinuano per accedere con maggiore facilità nella nostra Nazione e all'interno della nostra società. Per questo la vigilanza attenta e scrupolosa è la migliore garanzia, sia per i cittadini italiani che per quelli ucraini. signor Presidente, lo spirito del decreto-legge in esame appare coerente con i valori e i principi che tutto il centrodestra ha sempre propugnato: solidarietà, assistenza, vigilanza. Ritengo che sia un testo da condividere e sarebbe un bel segnale se anche le opposizioni, spogliate della loro funzione istituzionale di opposizione parlamentare, decidessero di condividerne lo spirito e il merito.

Da più di un anno ci troviamo di fronte a un evento di politica internazionale che ha sconvolto la scena globale, ha riportato molto indietro le lancette dell'orologio e suscitato inquietudini diffuse e soprattutto grandissime sofferenze in uno dei Paesi del nostro Continente. La guerra è tornata in Europa con il suo il suo volto peggiore, sotto forma di invasione da parte di una Nazione con un Governo autoritario ai danni di un Paese indipendente da più di trent'anni, geloso della propria libertà e che cerca di difendere il proprio diritto ad essere un'entità politica integra e autonoma. Purtroppo, le incognite sono ancora molte. Continua a scorrere il sangue e continuano ad esserci morti, bombardamenti, violenze, torture. Apprendiamo in continuazione notizie che ci straziano e che spezzano i nostri cuori. La comunità internazionale, di fronte a un evento così eccezionale e straordinario, è chiamata a mettere in campo una reazione adeguata adeguata sotto tutti i punti di vista. Per fortuna, l'Europa e l'Occidente non hanno avuto, tranne rarissime eccezioni, esitazione alcuna nel fornire sostegno al Paese aggredito, alla sua popolazione così massicciamente minacciata dall'aggressività dell'invasore, alle persone più deboli che si sono ritrovate improvvisamente senza una casa, in difficoltà a reperire l'essenziale per il soddisfacimento delle necessità più elementari, in continuo pericolo di vita e a rischio in tutti i sensi. Lo hanno fatto con grande determinazione, con uno sforzo concertato. Il nostro Paese ha fatto la sua parte, ha dato il suo contributo e, come sappiamo, il sostegno a tante forme, quello più immediatamente necessario del sostegno militare per resistere all'aggressione. Ma c'è stata anche una grandissima mobilitazione sul piano umanitario e dell'accoglienza: proprio questo questo decreto-legge, che per fortuna ha visto unite le forze politiche e che cerca di provvedere a tutti i mezzi che sono necessari per far sì che lo sforzo di accoglienza sia sia razionale, ordinato, efficace e che abbia gli strumenti legislativi per conseguire rapidamente i propri scopi e possa ottenere i risultati che tutti ci attendiamo finché l'emergenza durerà. Servono risorse finanziarie e possibilità, per chi deve prendere decisioni, di prenderle rapidamente e con effetto immediato. Serve, insomma, avere tutta una serie di strumenti che ci permettano di rispondere a un'emergenza che - lo ripeto - ha sconvolto il nostro Paese e le opinioni pubbliche di tutto il Continente europeo e rappresenta un elemento imprescindibile per chiunque voglia dare affermazione concreta ai valori di solidarietà e di umanità. Ovviamente, in questo sforzo i poteri pubblici non sono soli. Come spesso accade, nel nostro Paese possiamo contare su una rete di associazionismo, di volontariato, di persone che disinteressatamente si mettono a disposizione di chi ha più bisogno, che riesce a moltiplicare

delle minacce più terribili che abbiamo visto sul suolo europeo negli ultimi decenni. il provvedimento che ci apprestiamo a votare è ovviamente un provvedimento *bipartisan*, come dimostrano gli interventi che mi hanno preceduto.

è facile essere strumentalizzati quando si è dall'altra parte della barricata, quando si è all'opposizione. È più difficile, però, mantenere poi la parola quando si è al Governo del Paese. Questo Governo lo sta dimostrando. Oggi Governo e Parlamento sono uniti nella difesa di un popolo che è soggiogato da una guerra ingiusta. Non entriamo nel merito della questione relativa allo stanziamento delle armi, perché non è questo l'oggetto del provvedimento è giusto ricordare che il Governo lavora per la pace dell'Ucraina. Se non ci fossero state quelle armi, l'Ucraina sarebbe stata occupata nel giro di dieci giorni dalla Russia. Quindi, noi questo lo dobbiamo a quel popolo che soffre tutti i giorni. Per venire alle misure che stanzia il decreto, sono misure molto tecniche. Tra queste, ad esempio, c'è una misura straordinaria ed eccezionale, che deroga alle altre già esistenti in materia di profughi. È la protezione temporanea,

di godere dei diritti civili fondamentali di cui godono i cittadini italiani. Possono addirittura lavorare e avere l'assistenza sanitaria dei nostri concittadini. Chi ne ha diritto? Hanno diritto alla protezione temporanea tutti i cittadini ucraini che abbiano maturato la residenza nel loro Paese a far data entro il 24 febbraio 2022 e così anche i loro familiari.

Con la norma in esame si prorogano anche i permessi di soggiorno, che vengono rilasciati dalla questura competente per territorio fino alla data del 31 Vi è una norma ancora più interessante in questo decreto, che ha valenza ancora più eccezionale, che è quella dell'articolo 2-*bis*. Essa coglie due aspetti fondamentali: intanto, dona dignità ai cittadini ucraini, che possono lavorare sul nostro territorio esercitando la professione medica e sanitaria; modo, consente anche ai nostri ospedali e alle nostre strutture pubbliche di alleviare la lacuna di personale. Come saprete meglio di me, l'Ucraina non ha albi professionali. A queste persone, che sono professionisti al pari dei nostri medici, nostri medici, basta una dichiarazione resa in tribunale, asseverata, per consentire loro di espletare la loro attività in Italia. È una procedura semplificata, appunto, che ci fa comprendere quanto il Governo sia vicino a queste persone, non solo in tema di accoglienza, ma anche nella volontà di una loro integrazione sul territorio nazionale. L'articolo 3 stanzia, inoltre, importanti risorse per i minori non accompagnati, che spesso sono le vere vittime in un conflitto come quello che stiamo vivendo in questo lungo anno. risorse che vengono affidate agli enti locali, per circa 40 milioni di euro, e che sono destinate alla cura dei bambini non più sotto forma di rimborso, come era previsto prima, ma di contributo, nella misura di 100 euro *pro capite*. È ovvio che un afflusso così cospicuo di persone necessiti anche di una risposta da parte dell'amministrazione dello Stato con l'assunzione di nuovo personale. Così il decreto prevede l'assunzione di nuove 10 unità, che vanno a rimpinguare la

40 milioni per gli enti locali e 232 milioni per il Viminale, per tutte le operazioni e le procedure di supporto ai profughi. Vorrei concludere il mio intervento intervento abbracciando idealmente il popolo ucraino. Credo che lo possiamo fare tutti e certamente questo è un pensiero condiviso da tutti.

Aspettiamo i ragazzi, le ragazze, gli uomini e le donne ucraine in Italia, come turisti in visita al nostro bel Paese, per abbracciarli finalmente da uomini liberi.

Signor Presidente, soltanto poche parole per associarmi ai colleghi che hanno manifestato, nel corso della discussione, la loro solidarietà e la loro vicinanza al popolo ucraino, che sta soffrendo un'aggressione che purtroppo non sembra avere termine. Abbiamo ogni giorno di fronte agli occhi immagini agghiaccianti: una popolazione indifesa, scuole e ospedali, insediamenti civili immagini agghiaccianti di sevizie e di crimini di guerra nei confronti di soldati e di civili. Ci sono purtroppo notizie che riguardano anche crimini nei confronti dei bambini. L'Italia, che è una grande democrazia, la Repubblica italiana è vicina al popolo ucraino, è vicina ai profughi ed è vicina a coloro che sono scappati dalla guerra e si sono rifugiati in tutti i Paesi europei e anche in Italia. Credo che oggi noi facciamo il nostro dovere di solidarietà nei confronti di un popolo europeo e di un popolo fratello che sta subendo una guerra ingiusta. Non posso che associarmi a tutti coloro che auspicano e hanno auspicato anche oggi che questa guerra possa avere termine e che la Russia ritiri le sue truppe e cessi questa aggressione. *(Applausi)*.

gli onorevoli senatori che hanno contribuito a svolgere un lavoro importante per portare a termine l'esame di questo decreto-legge.

4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, nonché inammissibile l'emendamento 3.1. Passiamo all'esame

Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, a oltre un anno dall'invasione russa nei confronti dell'Ucraina, il tema della guerra è purtroppo ancora all'ordine del giorno e più attuale che mai,

ringrazio, Presidente, anche perché ribadisco che è abbastanza emozionante parlare di bambini trucidati e ammazzati e anche di soldati ai quali è stata mozzata la testa. Nonostante la ferma e decisa controffensiva attuata dalle forze militari ucraine, l'esercito russo colpisce ancora senza sosta, non più - appunto - solo obiettivi militari, ma anche quartieri residenziali, scuole, ospedali, chiese, bambini, militari inermi. Prima di entrare nel merito del decreto-legge del quale ci apprestiamo oggi alla conversione, è doveroso fare alcune brevi considerazioni politiche. Grazie, Presidente, la sensibilità nei confronti della guerra dovrebbe essere di diverso genere. Il 24 febbraio dello scorso anno non è stato solo l'inizio di un'inaccettabile guerra di confine: con l'invasione delle forze militari di Mosca su un territorio sovrano e riconosciuto da tutta la comunità internazionale, si è rotto un equilibrio. È una rottura a cui tutti noi dobbiamo opporci sottolineando le atrocità non solo sotto il profilo geopolitico che questo conflitto comporta, ma ancor prima sotto l'aspetto umanitario, che è e deve rimanere il nostro primo pensiero. Ecco perché è fondamentale ribadire ancora una volta il sostegno dell'Italia all'Ucraina con tutte le nostre forze disponibili; un sostegno e un supporto che il presidente del Consiglio Meloni e tutti i Ministri dell'Esecutivo non hanno mai fatto mancare in questi mesi. Ecco perché il Governo ha sempre avuto una posizione chiara e decisa sulla gravità che emerge in tutta la sua profondità in queste ore e soprattutto sulla responsabilità dell'invasione russa in Ucraina, nonostante il ministro degli esteri russo Lavrov in questo momento stia dicendo che vuole addivenire a una pace. una pace. Ecco perché - ed è ancora più importante ricordarlo, colleghi - è doveroso sottolineare la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev dello scorso febbraio, ancora febbricitante, quando la *Premier* davanti a una fossa comune, quella di Buča, città simbolo della resistenza ucraina, ha deposto un mazzo di fiori tra le lacrime di tutti

La guerra che l'Europa sta vivendo è tuttavia anche un dramma umanitario che non può lasciarci indifferenti; un dramma umanitario che penso abbia colpito tutti noi, ognuno di noi in quest'Aula, ogni rappresentante del Governo.

In caso contrario, si avrà l'impressione che qualcuno, oltre a una vicinanza di facciata, non abbia il coraggio e la volontà di sostenere con forza la popolazione ucraina, lasciando solo il nostro Paese a livello internazionale e - cosa forse ancora più grave - il popolo di quella Nazione. Oggi l'Italia riveste un ruolo fondamentale sullo scenario politico internazionale. Questo ruolo da protagonista non è certo mancato sotto il profilo della solidarietà e della vicinanza alla popolazione e non mancherà in futuro. Siamo stati sin da subito tutti protagonisti per quanto concerne gli aiuti umanitari e l'accoglienza ai cittadini in fuga e il decreto-legge oggi oggetto della nostra discussione ne è l'ennesima prova. Non è certo un caso quindi che - secondo i dati dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, come è stato citato più volte durante questi minuti - l'Italia abbia accolto già più di 170.000 profughi dall'Ucraina. È un dato significativo che prova come gli attacchi di una certa opposizione che vuole screditare la nostra Nazione a livello internazionale, oltre che essere palesemente ideologici, sono soprattutto falsi e sbagliati. È inutile negarlo: più qualcuno dice che l'Italia viene isolata nei contesti geopolitici internazionali e più l'Italia, al contrario, con il nuovo Esecutivo guidato dal *premier* Meloni, svolge un ruolo sempre più da protagonista in Europa e nel mondo intero. Ieri il «Wall Street Journal» ha definito il *premier* Meloni autorevolissimo. Siamo fortemente convinti della necessità di dover affrontare la conversione in legge di questo decreto-legge per la protezione temporanea delle persone provenienti dall'Ucraina - come detto precedentemente - non abbiamo timore a sottolineare che questo Governo non solo si impegna sotto il profilo politico, ma si adopera anche con convinzione e concretezza per far fronte alla grave crisi umanitaria che sta attualmente colpendo l'Ucraina. Come è noto, tale crisi ha portato ad una massiccia ondata di sfollati e rifugiati che da mesi cercano protezione e assistenza all'estero. La situazione è estremamente critica e pertanto richiede una risposta urgente e coordinata da parte della comunità internazionale. Ogni Paese deve attivarsi in questa direzione. L'Italia ha fatto sin da subito la propria parte e continuerà a farla affinché possa essere fornita una protezione temporanea per i cittadini ucraini che si trovano in Italia; una protezione fondamentale che consentirà loro di rimanere nel nostro Paese, seppur per un tempo limitato, nel quale potranno ricevere assistenza medica, sociale e legale. il compito del nostro Paese non è solo l'accoglienza, ma anche e soprattutto l'integrazione. Mi permetta, Presidente, di fare riferimento e di ringraziare, come è stato fatto poc'anzi, tanti amministratori locali. Penso ad esempio ai mille che, con le difficoltà di ogni giorno, hanno dedicato e dedicano ancora oggi parte del loro tempo prezioso a migliorare la sinergia tra le comunità ucraine e le nostre realtà locali. È una sinergia che funziona e, proprio per questo, deve essere in misura ancora maggiore compito della nostra Nazione garantire a tutti i diritti di chi fugge veramente, ma solo veramente dalla guerra. È fondamentale dare il primo supporto alle persone che si trovano in situazioni di difficoltà. L'ambasciatore dell'Ucraina in Italia Melnyk, recentemente sollecitato sull'atteggiamento delle istituzioni italiane, ha detto testualmente che sono profondamente grati all'Italia per quello che ha fatto, per quello che sta facendo e per quello che farà in futuro. futuro. È una testimonianza simbolica che ci fa comprendere quanto sia apprezzato il lavoro che stiamo facendo. Importante è anche la testimonianza di un'associazione culturale italo-ucraina che ricordo essere della provincia di Brescia che si chiama Nadiya, che che in ucraino vuol dire speranza, che, nata nel 2002, da sempre opera per l'integrazione della comunità ucraina in Italia, in collaborazione con le istituzioni locali. All'indomani del conflitto dello scorso anno ha organizzato assistenza ai rifugiati su vari territori e li ha supportati con corsi di italiano per integrarsi meglio con la popolazione locale. Oggi quei rifugiati, sollecitati nella possibilità di un rientro a casa, hanno risposto - con nostro grande orgoglio - che la loro casa è l'Italia! Presidente, la presenza in Italia dei profughi ucraini esisteva già in parte prima del conflitto dello scorso febbraio, sia per le tante donne che accudiscono le nostre case, che già fuggivano dalla povertà, sia perché molti cittadini si erano da tempo mobilitati per lasciare la propria terra in seguito a insostenibili tensioni e conflitti etnici sul proprio territorio. La situazione è ovviamente peggiorata con l'inizio dell'invasione e dell'occupazione in gran parte del territorio e - secondo il già citato Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'organo più autorevole in materia - circa 8 milioni di persone sono state colpite dal conflitto, compresi gli oltre 2,8 milioni di sfollati interni e circa 2 milioni di rifugiati, o forse molti di più, che hanno cercato protezione all'estero. Diversi Paesi hanno adottato politiche per l'accoglienza dei rifugiati ucraini in seguito all'invasione, fra cui la Polonia, Paese che spesso è stato oggetto di critiche, anche in queste Aule, ma che oggi ha dato a tutta l'Europa una grandissima lezione di umanità. Concludo, Presidente, riportando alcune parole dette a margine dell'importante visita del presidente Meloni a Kiev al presidente Zelensky: chi sostiene, anche militarmente, l'Ucraina è chi lavora per la pace. Sono certa che converrete tutti con me nel ritenere che dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare ogni cittadino ucraino in difficolta con ogni mezzo, purtroppo.

Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della nostra componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto - esattamente come è avvenuto alla Camera alcune settimane fa - su questo provvedimento,

ovviamente, il nostro voto favorevole non mancherà. Si tratta di persone che scappano dalla guerra, persone che soffrono e, quindi, come è del tutto evidente - ripeto - non faremo mancare il nostro supporto. Mi limiterò semplicemente in questi minuti a

Diamo una mano a un popolo che soffre per una ingiustificabile e ingiustificata aggressione, lo sosteniamo in tutti i modi, mettiamo delle risorse a sua disposizione cercando però di fermare quella corsa agli armamenti - addirittura anche simbolicamente - che, purtroppo, ha caratterizzato e sta caratterizzando lungamente questa stagione politica. Questa è una stagione politica

se questo dovere morale e politico lo sentissimo sempre, quando parliamo di tutte le guerre che attraversano il mondo.

penso sia molto meno giusto invece non avere adeguate politiche di accoglienza nei confronti di chi scappa da guerre più lontane, magari da Paesi di cui a stento conosciamo il nome. Avremo ovviamente tutto il tempo di parlarne

A proposito di accoglienza, stiamo discutendo di un decreto molto importante, il cosiddetto decreto Cutro, sul quale stiamo registrando anche degli elementi di dissenso molto forti tra la maggioranza e la minoranza. È un decreto-legge fondato, per l'appunto, sul tema dell'accoglienza e

anche ad altre situazioni, faremmo una cosa molto giusta. Penso invece che l'abbassamento della soglia di attenzione e le scelte politiche che poi si fanno - per esempio, quando si parla di blocco navale, per lasciare la gente in mezzo al mare, gente che anche in quel caso scappa dalle guerre, esattamente come scappa dalla guerra in Ucraina

in esame, non è inerente all'accoglienza, ma ha a che fare con quello di cui stiamo discutendo oggi. C'è un nesso tra la situazione della guerra in Ucraina e le politiche di accoglienza che mettiamo in campo per dare qualche elemento di tutela ai profughi che arrivano. Allora, signor Presidente, quando facciamo un bilancio serio su questo primo anno di guerra?

favorendo una fine rapida della guerra? O sono scelte politiche e militari che rischiano di allungare la guerra ancora di più

di persone. Non voglio utilizzare questi minuti per dire una cosa che peraltro il mio Gruppo parlamentare e il mio partito stanno dicendo da più di un anno, opponendosi all'invio delle armi, com'è noto. Non voglio utilizzare questi minuti per discutere di questo. Penso però che tracciare un bilancio su come l'aver puntato solo ed esclusivamente sull'invio delle armi, e aver quindi sostanzialmente ragionato molto poco su quali possibili iniziative diplomatiche costruire per arrivare rapidamente, o comunque il più rapidamente possibile, alla cessazione della guerra e quindi anche evitare i suoi effetti più drammatici, sia una questione che dovremmo avere sempre la forza di affrontare e di cui dovremmo discutere. Altrimenti c'è un grande rimosso: è come se ci fosse una omissione di ragionamento, è come se discutessimo semplicemente degli effetti e non delle cause. Naturalmente non voglio essere frainteso: io ritengo che la causa principale sia l'aggressione di Putin all'Ucraina; aggressione che considero considero detestabile da tutti i punti di vista e, quindi, non mi sentirete mai esprimere una sola parola di distanza da questo; massima solidarietà all'Ucraina aggredita e sicuramente riconoscimento che la causa principale del conflitto sta in questo. però che un bilancio più serio su quello che è accaduto in questo anno e anche sull'assenza dell'Europa come soggetto politico che avrebbe dovuto farsi carico di una possibile strada diplomatica

riconosciuto che non c'è possibilità alcuna che la guerra finisca in maniera militare, e cioè con la vittoria militare di una parte nei confronti dell'altra. È evidente

un effetto di queste scelte dal mio punto di vista molto poco condivisibili. Vorrei semplicemente dire che il nostro voto a favore del provvedimento in esame non significa però mettere da parte tutto ciò che abbiamo cercato di dire

l'azione e la posizione del Governo attuale e di quello precedentemente per ciò che concerne la crisi in Ucraina; e questo sia quando si è trattato di prorogare l'autorizzazione a destinare mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative ucraine, sia a maggior ragione oggi, che ci troviamo a prorogare la disposizione che il Governo Draghi, prima dell'Esecutivo attuale, ha preso per proteggere le persone provenienti dall'Ucraina. Come ci è stato illustrato nel marzo del 2022, l'Unione europea ha attivato questo meccanismo, che è abbastanza unico nel suo genere e che non era mai stato attivato in precedenza. Questo ci restituisce anche la fotografia della gravità e dell'unicità di quanto sta avvenendo ormai da più di un anno in Ucraina e che, ahimè, solo parzialmente riusciamo a supportare come vorremmo. Si tratta di una forma eccezionale di protezione che garantisce immediata tutela a favore delle persone sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito dell'invasione da parte delle forze armate russe. Ribadisco che è bene ricordare anche a chi cerca di normalizzare - ahimè peraltro l'opinione pubblica, come in tutte le tragedie, un po' si abitua a tutto quello che accade - la gravità di quello che continua a succedere in Ucraina. Quindi, ricordiamoci sempre che questa procedura non era mai stata adottata in precedenza e lo è stata solo a seguito del richiamo dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, che ha invitato tutti i Paesi a consentire ai civili un accesso indiscriminato ai propri territori, e quindi a chiunque sia in fuga dalla guerra, come avviene con questo atto; ciò al di là delle normative nazionali, ma in rispetto dei generali principi di non respingimento, che sappiamo essere alla base della civile convivenza tra i Paesi europei, sullo *status* di rifugiati,

qualora dovessero sfuggire da tragedie come quelle di una guerra. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ribadisce tale principio. E lo dico per ricordare che quello di quello di accogliere quelle persone è un atto riconosciuto loro in quanto titolari di diritti. Tale misura fu recepita dal Governo Draghi - come è stato detto - il 28 marzo 2022, e a quel recepimento sono seguiti - è importanti richiamarlo anche al fine di darvi continuità - un piano nazionale e tutta una serie di atti governativi che hanno determinato la *governance* di tutti i processi che dipendevano da quel decreto-legge. Parliamo di un tema estremamente importante, di un dramma nel dramma che riguarda moltissime persone. Attualmente sono 4 milioni le persone che provengono dall'Ucraina e che beneficiano in Europa del meccanismo di protezione temporanea; in Italia sono quasi 174.000, secondo i numeri che ci sono stati consegnati il 17 febbraio 2023.

che ha visto distrutta la propria casa, che ha visto massacrata la propria città, che ha visto morire i propri cari, che ha dovuto lasciare il proprio lavoro, le proprie tutele, la propria scuola (per chi studiava), il proprio mondo, la propria socialità. Con questo atto viene concessa di fatto, per il tempo in cui l'Unione europea dà questa indicazione, tutta una serie di diritti che sono sì temporanei, ma hanno una limitazione solo nel tempo, perché dal punto di vista della profondità della normativa dovrebbero equiparare in tutto e per tutto la persona che viene accolta al cittadino italiano. Si hanno un titolo di soggiorno che consente di soggiornare regolarmente all'interno del territorio dello Stato; il diritto di esercitare qualsiasi attività di lavoro, subordinato o autonomo; il diritto di partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione professionale per gli adulti e per i più giovani; il diritto di essere integrati e inseriti nelle scuole; il diritto di essere adeguatamente alloggiati e di ricevere, se necessario, i mezzi per ottenere un'abitazione, nonché l'aiuto necessario in termini di assistenza sociale, assistenza sanitaria, cure mediche e di accedere a tutti i percorsi - già l'ho accennato - relativi al sistema educativo e alla tutela dei minori. Questo in linea di principio è stato affermato ed è nel nostro ordinamento. In questo anno è stato complesso declinare in tutti gli aspetti operativi questo diritto. Oggi il meccanismo è abbastanza oliato e consolidato sui vari punti. Ci sono ancora però criticità, ad esempio rispetto alle ASL, anche se, dal punto di vista del diritto, con il permesso di soggiorno per protezione temporanea è garantita l'assistenza sanitaria in Italia con le stesse tutele garantite ai cittadini italiani. Basterebbe recarsi presso una ASL per avere l'assegnazione del medico di medicina generale e di un pediatra a scelta, e ricevere poi tutte le prestazioni conseguenti. Questo meccanismo in alcune aree del Paese ha funzionato molto bene, in altre aree non ha funzionato con lo stesso automatismo. Anche se il codice STP per stranieri

dal precedente Governo sono state definite procedure per l'attivazione di questi *iter* da parte dei centri per l'impiego. Se in questa discussione posso sollecitare il Governo su un aspetto, vorrei dire che alcune criticità, già insite nelle procedure di accompagnamento e di riferimento nel mondo del lavoro dei cittadini italiani eseguite dai centri dell'impiego, ahimè, in virtù di questo-legge sono emerse anche per le persone accolte, soprattutto per la parte che riguarda la mappatura delle competenze, la ricostruzione dell'abilità e la possibilità di inserire in un percorso formativo le persone che scappano dall'Ucraina e vengono accolte da noi. Questo decreto non può che vederci d'accordo. Tutto ciò che viene fatto per supportare il popolo ucraino in questa tragica guerra è da noi visto con il massimo sostegno. Tuttavia, sempre per restare ad alcune criticità ed ambiti di miglioramento di questa norma, vi sono alcuni aspetti che possono e pensavamo potessero essere migliorati. Ad esempio, sono emerse alcune criticità con riferimento alla platea di coloro che possono essere destinatari dell'intervento di accoglienza secondo questa norma. Di fatto, la normativa italiana è in qualche modo più restrittiva di quella europea sotto alcuni aspetti. non prevede l'applicazione della protezione temporanea ad una serie di casi, che non sono però così esigui, come il caso di cittadini di Stato terzo che soggiornavano in Ucraina in modo regolare, in forma di un permesso di soggiorno, ma non permanente. ove fossero state in fuga e ce ne fossero state molte, non avrebbero il diritto al permesso; così come non lo hanno i cittadini di Stati terzo apolidi che soggiornavano irregolarmente in Ucraina oggi non avrebbero riconosciuto alcuno dei possibili strumenti di accoglienza che abbiamo sottolineato per i cittadini ucraini. La mancata inclusione dei soggetti che ho illustrato - ed ho portato soltanto alcuni esempi - si traduce, di fatto, in una forma di protezione selettiva, che lascia privo di tutela un numero rilevante di persone. Per questo invitiamo il Governo a valutare, anche con provvedimenti successivi, delle modalità per non escludere questi soggetti o comunque a trovare il modo di accoglierli e dare loro le tutele cui hanno diritto. Concludo, signor Presidente e colleghi, con una riflessione. Sono sicura che la discussione di oggi, che ci ha visto concordi sia alla discussione generale che alla presentazione di emendamenti, anche se con qualche distinguo e con qualche correttivo - sia stata utile per migliorare le norme presenti nel decreto e per limare alcune criticità. Non posso immaginare che in quest'Aula vi sia ancora qualcuno che non ritenga di dover accogliere chi scappa dalla guerra in Ucraina. Voglio, però, dire una cosa, a costo di sembrare evidente che vi sia un macro tema, il cosiddetto "elefante nella stanza", che non si può eludere: non possiamo parlare di accogliere le persone che fuggono dalla guerra in Ucraina senza parlare di nuovo della guerra in Ucraina. Ne abbiamo già parlato in quest'Aula più volte, ma è un tema che vede anche posizioni diverse, come abbiamo sentito poc'anzi da parte di alcuni colleghi. Noi abbiamo detto e abbiamo ribadito che, pur nel nostro ruolo di opposizione, il Governo ha il pieno supporto del Gruppo Azione-Italia Viva per quanto riguarda il sostegno militare all'Ucraina, affinché possa difendersi dall'aggressione russa. Non possiamo, però, parlare di accoglienza senza ricordare che esiste un tema accoglienza perché esiste un tema guerra. Non possiamo oggi fare una discussione edulcorata, dicendo che dobbiamo accogliere tutti coloro che scappano dalla guerra - e ci mancherebbe altro - senza ricordare che il principale motivo per cui oggi vi sono rifugiati è che, ancora prima di essere quello ucraino un popolo

la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2023, che ci dice che non c'è tanto ottimismo sulla cessazione prossima del conflitto e che, anzi, l'analisi degli accadimenti più recenti suggerisce una prognosi molto lunga. È un dato sconfortante, perché la guerra che da febbraio 2022 sta sconvolgendo l'Ucraina è destinata a durare, con il suo carico di tragiche conseguenze di morte e di fuga, spingendo milioni di persone a fuggire da quel Paese. tra gli Stati più esposti a questo fenomeno, sono moltissime le persone già arrivate nel nostro Paese che dobbiamo accogliere con la massima solidarietà, attesa la loro fragilità e la loro debolezza. Per questo mi auguro il massimo consenso possibile da parte dell'Assemblea del Senato. Allo stesso tempo, il dato di una proroga, che lascia presagire un conflitto molto lungo, deve essere letto anche nell'ottica di tributare grande merito all'orgoglio di un popolo fiero e combattivo come quello ucraino. La resistenza indomita dell'Ucraina, la sua determinazione e la sua fierezza hanno dimostrato che non era ovvia quella vittoria lampo che appariva al Cremlino. Non era ovvia anche alla luce del fatto che la parte più civile del mondo ha boicottato la Russia, considerato che il sostegno militare occidentale si è rivelato decisivo. Non mi sento un guerrafondaio e non me ne vogliano quelle forze politiche che più criticano l'aiuto militare; ma cosa sarebbe accaduto se la civiltà occidentale non avesse dimostrato quella prontezza di soccorso altruistico, anche sul piano tecnologico e sul piano degli armamenti? Cosa sarebbe successo per quel popolo? Cosa sarebbe successo per noi e per la nostra sicurezza futura? Ciò detto, rimane la doverosità di uno sforzo ulteriore per la pace, che non può essere ottenuta con la resa; questo è inaccettabile. Il disegno di legge che oggi discutiamo ha una fonte molto remota, una direttiva europea del 2001, che è stata recepita nel nostro ordinamento nel 2003 e che prevedeva la protezione temporanea in caso di esodi di massa, con l'obiettivo di una tutela comune europea, tutela mai attivata prima del conflitto ucraino. Si è sempre sperato in una direttiva che non si dovesse mai attivare, quasi come fosse una clausola di stile, e invece è ormai più di un anno che essa caratterizza gran parte della vita istituzionale dei Paesi europei. Il nostro presidente Berlusconi, a cui va il mio e il nostro affetto, che salutiamo e che è prossimo a una guarigione totale *(Applausi)*, ha sempre sostenuto che l'Europa dovrebbe dotarsi non solo di una sola politica estera, ma di un esercito e di una difesa comune, con un ruolo forte e integrato nell'Alleanza atlantica. Non esisteva e non esiste, in nessuna guerra, un lato positivo; esistono però degli effetti indiretti utili. Il conflitto infatti ha accelerato la transizione ecologica nel nostro Paese e il percorso della sua indipendenza energetica. Qui noi non dovremmo fare battaglie di retroguardia, ma dovremmo pensare al futuro con uno sguardo legato anche a a una transizione verde, non solo del nostro Paese, ma della nostra economia, che può porci in vantaggio rispetto alle altre Nazioni europee. Ciò ci deve essere anche di monito: non dovremmo aspettare le tragedie per adeguare il nostro ordinamento agli schemi istituzionali più moderni e più efficienti. Penso al ponte Morandi e ad alcune innovazioni normative oggi confluite nel nuovo codice degli appalti. Penso al Covid e ad alcune semplificazioni amministrative nell'accesso al pubblico impiego, oggi confluite in provvedimenti più generali. In tal senso auspico un percorso di riforme più ordinato e programmato, figlio di una visione non giustizialista e legata alla semplificazione procedurale, a cui il Paese ha dato il proprio consenso democratico. È un'ottima cosa per noi garantire l'assistenza ai rifugiati ucraini all'ingresso del nostro Paese, anche quando i flussi di accesso risultano incompatibili con il sistema di solidarietà ordinario, sostenendo anche soluzioni di assistenza temporanea sussidiaria in grado di garantire sostegno in attesa dell'inserimento nel sistema di accoglienza ordinario e istituzionale. essere un popolo che ospita, cioè che dà un posto e non solo un posto qualunque, ma un posto d'onore a chi viene per la guerra, a chi viene per la miseria, a chi fugge da queste disgrazie. È nel nostro DNA di italiani: abbiamo sempre avuto questa caratteristica tendenza all'accoglienza e alla solidarietà. Spero che tutto ciò possa a breve essere solo un ricordo, ma oggi è il tempo della responsabilità e della solidarietà. Oggi è il momento nel quale dobbiamo fare i conti con le tragedie umane, ma anche quello nel quale farsi trovare maggiormente pronti per dare un ristoro a quelle vite sospese che attendono la pace. Una tragedia ancora più amplificata dalle barbarie del gruppo Wagner. Alcuni comportamenti disumani utilizzati da parte delle forze armate russe, colpendo bersagli e infrastrutture civili, colpendo abitazioni civili, già rendevano crudele e sproporzionata l'aggressione; ma l'eccidio di bambini è davvero intollerabile. Mi rifaccio alle parole del nostro Presidente della Repubblica, secondo due direttrici. La prima: l'Italia deve continuare a dare «sostegno all'Ucraina finché è necessario, finché occorre, sotto ogni profilo: di forniture militari, finanziario, umanitario, per la ricostruzione del Paese. Questo con la convinzione che ciò riguardi non solo l'Ucraina», ma, come ho detto prima, tutti noi, per la nostra sicurezza, ma anche per il nostro spirito di accoglienza e di solidarietà. Il ministro Tajani ha ribadito poche ore fa l'impegno dell'Italia per la ricostruzione e per l'adesione all'Unione europea dell'Ucraina. La seconda direttrice, dettata dal Presidente della Repubblica: «Serve una nuova politica di asilo (...), superando le vecchie regole» che sono ormai antiquate. Citavo prima, in proposito, una direttiva europea del 2001. Il problema deve essere rivalutato come problema dell'Unione europea, perché solo l'Unione europea può farlo con un'azione davvero coordinata. Noi di Forza Italia siamo stati i primi a dirlo, da tanto tempo. L'Unione europea è nata per difendere la libertà e la democrazia e per offrire accoglienza e solidarietà. Per questo la coesione europea è importante, per l'attualità, ma soprattutto per le giovani generazioni. Il nostro è un partito che si ispira a questi valori, oltre che liberali, anche europeisti e alle radici cristiane.

mesi di guerra, oltre 300.000 morti, anche se non abbiamo ancora dati precisi, milioni di profughi: sono cifre enormi, che non ci danno ancora, con esattezza, le dimensioni della tragedia che si sta consumando e di quello che sta succedendo in Ucraina. Credo che tutto il nostro popolo sia rimasto sconvolto da alcune notizie, come quella di ieri, sui due mercenari russi del gruppo Wagner, che hanno confessato di aver ucciso oltre 20 bambini e adolescenti ucraini. parole terribili, sentite pronunciare in un video: «Ho sparato alla testa di una bambina di cinque anni. Ho eseguito l'ordine con questa mano, ho ucciso i bambini, compresi bambini di cinque Hanno confessato anche l'esplosione di una fossa dove c'erano più di 50 prigionieri feriti e la pulizia etnica di alcuni edifici residenziali, uccidendo tutti, compresi i bambini. Sono sicuramente fatti terribili, che vanno oltre l'umanità. Quello che ci dovremmo chiedere è se stiamo facendo tutto il possibile per salvare quante più vite umane

Come possiamo pensare che questi atti possano non rimanere scolpiti nella storia della nostra umanità? Sentivo parlare il presidente del Consiglio Meloni, secondo cui dobbiamo perseguire una pace giusta, ma non ci sarà mai una pace giusta, perché quando vengono uccise centinaia di migliaia di persone, compresi i bambini, si creano cicatrici indelebili, che rimangono sulla pelle della civiltà umana. Queste situazioni rimarranno nella nostra storia e non ci sarà mai alcun modo per togliere l'odio da queste due popolazioni. Avremmo dovuto fare tutto il possibile per prevenire e mettere in atto tutte le misure diplomatiche per non arrivare a questa situazione.

Per noi la cosa più giusta è cercare di salvare quante più vite umane possibile. Questa è la cosa più giusta da fare. *(Applausi)*. Crediamo che non sia né giusto, né tollerabile che bambini di cinque anni vengano brutalmente uccisi, ferite che rimarranno per sempre nella storia della civiltà umana. Crediamo che non sia giusto non rispettare la nostra Costituzione, che prevede che l'Italia ripudi la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Avremmo potuto avere un altro ruolo, anche perché l'Ucraina non fa parte né della NATO, né dell'Unione europea, quindi il nostro aiuto al popolo ucraino poteva essere di altra natura.

e quindi il sostegno non può essere solo l'invio di armi. Crediamo che la cosa più giusta sia adoperarsi con tutti gli strumenti diplomatici possibili per evitare nuove vittime e per evitare un'*escalation* militare del conflitto.

Occorre capovolgere, quindi, la narrazione di una guerra dolorosa ma necessaria, perché abbiamo visto che non è così: questa guerra rischia di diventare pluriennale,

necessario parlare anche di un conflitto che è alle porte dell'Europa. Si parla ormai di armi nucleari tattiche in Bielorussia, che sono ordigni

È dunque possibile che ci sia un interesse collettivo europeo diverso da altri interessi? Forse si può dire, come ha fatto il presidente Macron, che l'interesse europeo è diverso da quello americano, a 8.000 chilometri di distanza dai campi di combattimento. Un ordigno nucleare in Europa coinvolgerebbe anche le nostre popolazioni, non quelle americane, quindi è possibile parlare di interessi europei diversi da quelli americani? Lo ha fatto il presidente Macron quando ha parlato di una strategia autonoma europea.

Hitler non aveva le armi nucleari, le forze in campo e le tecnologie belliche erano diverse, la storia è diversa, sono passati quasi ottant'anni, non possiamo non pensare che se Hitler avesse avuto un arsenale nucleare forse la Seconda guerra mondiale non sarebbe finita nello stesso modo. Dobbiamo pensare che questa è una guerra completamente diversa da quelle del passato, dobbiamo trovare gli strumenti diplomatici e metterli tutti in campo per cercare di alleggerire le tensioni. L'Italia poteva giocare un ruolo diverso rispetto agli altri Paesi, anche perché la sua Costituzione glielo consentiva. Oggi stiamo discutendo della conversione in legge di un decreto che dispone aiuti umanitari, accoglienza, protezione temporanea per i rifugiati ucraini. Vengono stanziate risorse importanti per alleviare i Comuni dalle problematiche derivanti dall'ingresso dei profughi ucraini per i centri di accoglienza governativi ordinari e straordinari. Vengono adottate misure importanti: viene prorogato il permesso di soggiorno agli ucraini che sono sul territorio nazionale e viene riconosciuta la qualifica professionale per il personale medico e sanitario sono misure importanti, ma, nello stesso tempo, pesano sul bilancio italiano per quasi 300 milioni di euro. Come si recuperano queste risorse? Attraverso tagli alla spesa sociale, agli ospedali, alla scuola

e, anche se questo comporterà un aggravio di spesa per lo Stato, noi la dobbiamo rispettare e dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare il popolo ucraino. Non dobbiamo però dimenticare che non è questa la soluzione, non è questa non è l'invio di armi che aiuta a non alimentare l'odio, anzi, fa il contrario. L'unica soluzione è fermare questa maledetta guerra ed esigiamo un cambio di passo del Governo, della NATO e dell'Unione europea lo stop all'invio di nuove armi. La pace è l'unica via possibile e l'Italia deve essere protagonista nell'avvio di un percorso diplomatico che porti alla pace.

noi diciamo convintamente sì a questo provvedimento, che purtroppo trae le sue origini da una terribile tragedia, ma che permette al nostro Paese di mostrare uno dei suoi lati migliori: il grande cuore della sua popolazione. L'accoglienza, la solidarietà e la generosità sono tratti distintivi della nostra gente, del nostro popolo, delle nostre comunità, che sanno aprire le braccia quando si trovano di fronte a persone che scappano dalla guerra, dalla morte, dalla distruzione della propria vita. Su questo dubbi non ce ne sono, perché il nostro Paese ha sempre dato prova di essere solidale e altruista con i profughi e in questo caso, a differenza di altre situazioni - checché se ne dica - abbiamo a che fare con veri profughi, con persone che abbandonano il proprio Paese perché davvero temono per la propria vita. Per questo credo che prima di tutto vadano ringraziati tutti quei Comuni, tutti quei sindaci e tutte quelle comunità che hanno immediatamente e senza tentennamenti dato la propria disponibilità per accogliere uomini, ma soprattutto famiglie, donne e bambini ucraini che scappano dalla guerra e lo hanno fatto nella consapevolezza che mai e poi mai il nostro Paese e il nostro popolo potrebbero dire di no a chi chiede aiuto; mai potrebbero girarsi dall'altra parte di fronte al dolore degli esuli che fuggono dall'aggressione russa. Con questo provvedimento mettiamo a disposizione una serie di misure per l'accoglienza: oggi si parla di circa 180.000 ucraini scappati dalle bombe e dalla morte per venire nel nostro Paese. Confermiamo il via libera alla protezione temporanea, una misura di carattere eccezionale dovuta alla gravità del momento, che permette di garantire a tutti i profughi una tutela immediata, senza il rischio di ingolfare il sistema d'asilo, visto che parliamo di veri profughi, ben diversi dai clandestini che in questi giorni sbarcano nel nostro Paese e che quindi avranno il diritto di ottenere asilo. Colleghi, la giornata di oggi può essere anche l'occasione per due ulteriori riflessioni che nascono da questo provvedimento, grazie al quale si capisce la necessità, proprio per reperire i fondi indispensabili a garantire un'accoglienza dignitosa a chi scappa dalla guerra, di fermare al più presto l'invasione di clandestini nel nostro Paese, contrastando la criminalità organizzata, i trafficanti di esseri umani e chi antepone il profitto e il *business* dell'accoglienza al diritto, alla dignità e alla vita degli stessi immigrati e il provvedimento che domani abbiamo in esame nell'Aula del Senato può rappresentare un'occasione. Infine, credo che la fuga di tante famiglie e di tanti bambini dall'inferno della guerra e del conflitto, la loro sofferenza e questa incredibile tragedia ci facciano capire l'importanza di di pronunciare un po' di più e un po' più spesso la parola "pace" rispetto alla parola "armi". Abbiamo un obbligo morale: porre fine al conflitto e non alimentare una pericolosa *escalation*. Per questo annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

mesi, non accenna a finire. Una guerra frutto di un'invasione dissennata da parte della Russia che ha provocato circa 5 milioni di rifugiati nei Paesi europei e 7 milioni di sfollati interni al Paese. Secondo i dati della Protezione civile, alla quale è affidata la gestione di questa emergenza, sono oltre 173.000 i rifugiati ucraini, come abbiamo già sentito, che hanno attraversato le nostre frontiere dal 24 febbraio 2022. Di questi, circa 169.000, 169.000, oltre il 98 per cento, hanno chiesto la protezione temporanea nel nostro Paese. È già stato osservato, ma è opportuno ricordarlo, che questa è la prima volta che è stata attivata la direttiva europea del 2001 che conferisce, cito testualmente: «protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati a cittadini non comunitari che non possono rientrare nel loro Paese, soprattutto a causa di guerre, violenze violenze e di violazione dei diritti umani». Non ci sono nel mondo purtroppo solo gli ucraini e su questo dovremo fare una seria riflessione. Dunque la stragrande maggioranza dei rifugiati ucraini hanno trovato ospitalità principalmente da amici e parenti e a loro a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Sono migliaia i nostri concittadini che hanno aiutato i profughi, aprendo le loro case, aiutato le loro famiglie, anche economicamente, inviando generi di conforto e partecipando a missioni di cooperazione. Grazie anche agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, ai ragazzi, che hanno accolto accolto con generosità i ragazzi ucraini, facendoli sentire assolutamente i benvenuti in tutte le scuole. Pochi hanno trovato ospitalità presso i centri di accoglienza straordinaria (CAS) o negli alberghi. Lo Stato italiano - e lo voglio sottolineare con forza per coloro che hanno scelto di non entrare nel circuito pubblico di accoglienza, ha dato un contributo annuo *una tantum* di 900 euro, poco più di 75 euro al mese, una somma davvero misera se si considera che molti di loro hanno con sé bambini e anziani. La cosa ancora più sorprendente è che il Governo ha pensato bene di coprire la spesa complessiva di questo decreto-legge, pari a circa 300 milioni di euro, togliendoli ad altri Ministeri, in particolare penalizzando il capitolo relativo alla cooperazione e allo sviluppo; un capolavoro di ipocrisia visto che, da mesi e mesi, la *premier* Meloni e i suoi Ministri ci parlano del cosiddetto piano Mattei. Sono mesi, dalla campagna elettorale di agosto, che sentiamo parlare del Piano straordinario per l'Africa; da un lato, dunque, si afferma che solo attraverso un piano straordinario di cooperazione con alcuni Paesi africani, potremo garantire all'Italia nuove fonti di energia tramite la stipula di accordi con Paesi come la Libia o l'Algeria e, dall'altro lato, si tolgono soldi alla cooperazione internazionale che, quelli sì, garantirebbero uno sviluppo sociale ed economico ai Paesi africani. Insomma un capolavoro di incoerenza, tenuto conto che quello di cui si parla, il piano Mattei appunto, è una scatola vuota per il momento, di cui non si sa assolutamente nulla, di cui non esiste nemmeno una *slide*, ma del quale la presidente Meloni continua a ripetere ogni giorno la grandezza e la necessità. Belle parole, senza alcun fondamento. Sarebbe ora di finire con la propaganda e cambiare registro, ma nonostante evidenti lacune e contraddizioni il Partito Democratico darà un sì convinto convinto a questo provvedimento, anche se la maggioranza è rimasta come sempre del tutto sorda alle nostre osservazioni e richieste di buon senso. Un sì convinto perché l'Italia si è da subito stretta, insieme all'intera Europa, accanto all'Ucraina, sostenendola in ogni modo, anche nella sua legittima difesa. Il popolo ucraino è vittima di un'assurda e spietata invasione da parte di un altro Stato e bene abbiamo fatto a stare al suo fianco e bene facciamo ad aiutare le persone che fuggono da una guerra tremenda. Voteremo sì perché c'è ancora bisogno, dopo più di un anno, di solidarietà concreta nei confronti dei cittadini ucraini che sono venuti e continueranno a venire in Italia per mettere se stessi e le loro famiglie al riparo dalla guerra. Sta a noi garantire la loro sicurezza.

dall'Ucraina è un atto dovuto che la nostra Nazione sente di indispensabile umanità nei confronti di un intero popolo. massacrato da un criminale aggressore, Vladimir Putin, sostenuto da un Paese, la Repubblica Popolare di Cina, che, se lo volesse, con un solo gesto - lo sottolineo - potrebbe fermare il conflitto, arrestare i bombardamenti a tappeto e privare Mosca di qualsiasi mezzo per alimentare una guerra indegna dell'essere uomini. Al contrario, il presidente Xi Jinping si guarda bene dal fermarla, ripeto, anche con un semplice gesto. Ascoltando le parole del relatore, senatore Balboni, gli interventi che mi hanno preceduto rileggendo i sei articoli del decreto-legge, compaiono qui in quest'Aula, dinanzi a noi, moltitudini di disperati, folle di disperati, feriti, con vestiti incredibilmente disastrati, case abbattute, enormi distruzioni. Abbiamo queste folle dinanzi agli occhi, occhi, le immagini di moltitudini di famiglie disperate, di donne e di bambini che vogliamo e dobbiamo assolutamente soccorrere appena essi arrivano nel rifugio sicuro, nel porto sicuro del nostro Paese e negli altri Paesi europei, europei, in un'Europa - per fortuna, ma non solo per fortuna - non ancora toccata dalle armi genocidarie di un aggressore che si chiama Vladimir Putin e dalle armi dei suoi complici. Le miriadi di fratelli ucraini che fuggono dall'Ucraina e che decidiamo di accogliere qui da noi avrebbero potuto rimanere nelle loro case; avrebbero potuto continuare a lavorare i loro campi e a produrre nelle loro grandi e piccole aziende. Avrebbero potuto e dovuto restare con i loro genitori le migliaia di bambini catturati e deportati dal Donbass e dalla Crimea in Russia da una mostruosa organizzazione guidata da una donna, che di donna ha tutto tranne che l'anima di madre. Una donna che nel disgustoso sistema putiniano viene qualificata come commissario per i diritti umani. avrebbero potuto continuare a vivere, a giocare, a crescere. Di quei bambini parlava stamane - è stato menzionato poco fa - un prigioniero dell'organizzazione terroristica russa Wagner;

i comandi che aveva ricevuto fossero tassativi. Erano comandi che il suo comandante aveva ricevuto da Prigozhin, il comandante del gruppo Wagner, che dicevano tassativamente: chiunque si incontri, qualsiasi civile, compresi i bambini, deve essere eliminato.

a sostegno del legittimo Governo di un grande Paese europeo aggredito da un regime farneticante. Ci vogliamo rendere conto, signor Presidente, - mi consenta di rivolgere questa domanda e questo appello anche a chi ha parlato prima di me, come il senatore De Cristofaro - che

oggi milioni di profughi e sfollati, centinaia di migliaia di vittime, migliaia di miliardi di euro di danni catastrofici? Le persone disperate che accogliamo in Italia sono

seppure in ritardo, essere fortemente aiutata e si deve fare di tutto affinché questa eroica Nazione sia così forte da poter vivere in pace nei suoi confini, intatti, nella cultura e nella democrazia alla quale essa dimostra di credere. Per questo motivo e per il forte significato che questo provvedimento di conversione di decreto-legge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

deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione. Giovedì 20